Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza di questa Assemblea fatti gravi avvenuti in provincia di Caserta e precisamente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere.

concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa d'asta, falso ideologico e appalti illeciti. Lo scandalo, fra l'altro, è stato scoperto grazie a un'intercettazione telefonica, che proprio il Governo Renzi vuole fortemente limitare. Chi è coinvolto in questo scandalo, signor Presidente, signori colleghi, che capisco bene non volete ascoltare perché duole all'orecchio ascoltare certe notizie? Il PD, coinvolto in questo scandalo, questa volta in Campania, ha propri esponenti indagati, Stefano Graziano, consigliere regionale della Regione Campania, Presidente del PD campano ed ex consigliere del Governo Letta e del Governo Renzi.

coloro che dovrebbero essere i nuovi senatori che comporranno il Senato della Repubblica così come voluto dal Governo Renzi, dalla ministra Boschi e dal senatore Verdini, con il suo Gruppo AL-A che ha votato questa riforma incostituzionale

fa, e si ponga davanti alle proprie responsabilità. Perché ricordo che questo è l'ennesimo scandalo, dopo Trivellopoli, che coinvolge, per l'ennesima volta, questo Governo. *(Applausi

La relatrice, senatrice Capacchione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

*relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il disegno di legge in esame, che riportiamo per la terza volta in quest'Aula, trae origine dalla necessità di arginare i comportamenti volti alla denigrazione a sfondo razziale, unitamente, talvolta, alla negazione tendenziosa di fatti storici riconosciuti. Esso pertanto è volto alla modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale è stata ratificata la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, introducendo il reato di negazionismo, cioè il divieto di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, ovvero di propaganda, di superiorità o odio razziale o incitamento a commettere reati di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, giunge quindi in terza lettura davanti a quest'Assemblea. necessario dare conto del fatto che l'*iter* parlamentare del testo in esame è stato molto articolato e per certi versi complesso, presso entrambi i rami del Parlamento, ciò a dimostrazione della difficoltà di un intervento normativo in una materia così delicata che sfiora diritti costituzionalmente garantiti, come le libertà di espressione e di opinione. In particolare, i lavori preparatori hanno evidenziato perplessità e criticità rispetto a quello che spesso viene appunto indicato come un reato di opinione che potrebbe limitare gli ambiti della ricerca storica o anche della libera espressione di un pensiero, sia pur odioso e repellente. Ricordo a quest'Assemblea che in prima lettura il Senato, con un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione, era giunto all'approvazione di un testo che qualificava come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, rispondendo all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione o di crimini violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero. Inoltre il Senato, modificando l'articolo 414 del codice penale, cioè l'istigazione a commettere dei reati, aveva previsto, al comma 2 dell'articolo unico del testo approvato, la riduzione del massimo di pena da cinque a tre anni per il reato di istigazione a commettere un delitto. In ragione dell'inopportunità di punire la negazione di fatti di genocidio con la stessa pena prevista per l'apologia, si era ritenuto d'intervenire sull'articolo 414 del codice penale anziché sulla cosiddetta legge Mancino. la Camera dei deputati ha soppresso le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e ha soppresso anche il comma 2, che modificava l'articolo 414 del codice penale; inoltre, ha aggiunto il capoverso 3-*bis*, in base al quale, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto «dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro». Tuttavia la Commissione, nell'ambito di un clima di condivisione tra tutte le forze politiche, ha ritenuto opportuno modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati,

al fine di poter circoscrivere il reato di negazionismo alle condotte che implichino il pericolo concreto di atti di discriminazione e, dunque, al fine di evitare il rischio di criminalizzare atti che possono essere espressione di libera manifestazione del pensiero. Quanto poi al riferimento a «i fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro», il dibattito in Commissione ha rilevato la forte ambiguità di tale formulazione, non tanto in ordine all'applicabilità dell'aggravante a fatti accertati in sentenze passate in giudicato, quanto per la difficoltà di ancorare tale applicabilità all'accertamento di fatti da parte di atti di organismi internazionali o sovranazionali dei quali l'Italia è componente. Anche sotto questo profilo, si è verificata un'ampia convergenza dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione per ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato. Quanto, poi, alla modifica all'articolo 414 del codice penale sulla riduzione della pena da cinque a tre anni, che pure era stata prevista dal Senato in prima lettura, la Commissione, alla fine, dopo un complesso ed articolato dibattito, ha deciso a maggioranza,

per evitare una distonia sistemica con la pena prevista al comma 4 del citato articolo 414 per i reati di terrorismo. In Commissione quindi, era stato proposto un emendamento (l'emendamento 1.23, che riformulava l'articolo 414 nel senso di dare coerenza al rapporto tra la fattispecie generale di pubblica istigazione, di cui al primo comma dell'articolo 414 del codice penale, e quella di cui al successivo quarto comma. Su tale emendamento mi sono rimessa alla Commissione, mentre il Governo ha invitato i proponenti al ritiro in vista di una più approfondita riflessione per questa Assemblea. I proponenti non hanno accolto tale invito e, con il parere contrario del Governo, tale emendamento è stato respinto. Infatti il Governo ha ravvisato che la riduzione di pena ivi prevista non appariva in sintonia con le previsioni edittali di pena per le fattispecie speciali di cui all'articolo 414-*bis* (istigazione a reati di pedofilia) e di cui all'articolo 415-*bis* del codice penale, entrambe punite, a fronte di una condotta di pubblica istigazione, con la reclusione nel massimo pari a cinque anni. Auspico che su questo punto l'Assemblea possa svolgere una meditata riflessione per giungere, alla fine, all'approvazione di un testo il più possibile condiviso.

Presidente, dovendosi procedere ad una votazione le chiedo di verificare preliminarmente

che negano in tutto o in parte la Shoah o altri crimini di genocidio, come riconosciuti dalla Corte penale internazionale, e quindi per un numero limitatissimo di casi. Sono passati

è bene mettere per iscritto nella nostra legge che quelle cose sono avvenute e che, al di là di una speculazione storica, che è sempre legittima anche quando demenziale, non è ammissibile e dunque è reato usare la negazione dello sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale sotto il regime nazista e altri regimi che collaborarono, tra i quali purtroppo quello che c'era nel nostro Paese, allo scopo di istigare all'odio. Si tratta di un disegno di legge estremamente equilibrato, che addirittura prevedeva la riduzione della

- la Camera l'aveva tolto, ma la Commissione giustizia l'ha nuovamente inserito - il requisito che tale istigazione, nel caso che interessa questa legge, con l'inclusione della negazione della Shoah,

disegno di legge è particolarmente importante in questo periodo? Perché c'è un aspetto storico. Quella generazione ormai, in gran parte, ci ha lasciati,

come quella di ieri, che dovrebbe unire gli italiani al di là del fatto che, come sappiamo bene, ricorda la fine di una guerra civile, dove alcuni italiani si schierarono da una parte e altri dall'altra. Ebbene, alcune celebrazioni i cui protagonisti sono i vincitori della guerra di liberazione, ovvero i membri della Resistenza, coloro che li aiutarono e - anche se parecchio dimenticati e messi da parte - quei 300.000 caduti di Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, India, Francia e tanti altri, che sono venuti a combattere

bene, dunque, che una legge lo ribadisca a chiare lettere: l'orrore di Auschwitz e dei tanti altri campi di sterminio, l'orrore che è avvenuto anche nel nostro Paese, nella nostra città, quell'orrore è stato e non può essere negato, e negarlo è un atto di violenza in sé.

furono approvate le leggi razziali, da molti giustamente definite leggi razziste (che sarebbe il termine più proprio), ed è pertanto molto appropriato che in queste stesse Aule si sancisca che quell'orrore è inaccettabile e che quell'orrore è stato e negarlo è inaccettabile. Lo dobbiamo per la verità storica, lo dobbiamo ai sopravvissuti, lo dobbiamo alla memoria dei tanti, dei milioni che furono uccisi e lo dobbiamo ai tanti che lottarono perché ciò non avvenisse mai più, italiani e non.

mi piace ricordare che nella scorsa legislatura il terzo firmatario fu la senatrice Rita Levi Montalcini, che quei fatti visse come testimone diretta, in quanto ebrea, fu esclusa da ogni possibile attività nel nostro Paese, insieme a tanti altri. Anche in memoria della nostra collega scomparsa,

Questo naturalmente suscita un problema: esiste uno specifico reato commesso da chiunque neghi la Shoah? Se così fosse, se questo fosse il contenuto del disegno di legge, avrei molte difficoltà a votarlo perché un signore, o uno studioso, che dica che non è vero che c'è stato lo sterminio degli ebrei, ma anche di molti Rom e di tanti comunisti, da parte dei nazisti è un cretino, è un signore che dice una evidente bugia

Esso si propone semplicemente di introdurre un'aggravante a reati già esistenti nel caso ci si riferisca a questo orrore assoluto, che è stato la Shoah.

anche storica su quel fatto che interroga tutte le nostre coscienze: c'è stato, è vero, è così, l'orrore è vissuto e si è dipanato nella nostra bella Europa, nella terra dei diritti. In secondo luogo, perché tale aggravante può servire per contrastare specifici reati. Qui si parla di istigazione a commettere reati contro l'umanità, non si parla di sostenere delle corbellerie. Chiunque sostenga corbellerie può essere criticato ma non portato in tribunale, chi invece sta istigando a commettere gravissimi reati può e deve essere portato in tribunale. Questa è la prima cosa da dire. La seconda considerazione che vorrei svolgere riprende

una prova di bestialità: è un fatto che nei campi di concentramento nazisti c'erano italiani ebrei, c'erano italiani comunisti, c'erano dei rom e che il nazismo si proponesse lo sterminio degli ebrei. Sono quindi vittime e già solo per questo avrebbero diritto ad essere presenti in prima fila nelle manifestazioni per il 25 aprile. Ma non è solo questo, perché alcuni ebrei, come alcuni cattolici e alcuni comunisti, hanno rischiato la vita per un futuro diverso della Repubblica, combattendo una guerra civile che non è stata facile da combattere e che è costata un prezzo anche personale e compiendo uno sforzo finale, intorno al 25 aprile, affinché le città italiane fossero liberate anche solo un giorno prima dagli italiani e non dagli alleati. Gli alleati avevano tutto il titolo per liberarle, ma la liberazione di Milano, di Torino o di Genova da parte degli italiani aveva un valore simbolico di grandissima importanza. secondo motivo fondamentale per chiedere alla Brigata ebraica di far parte delle manifestazioni per il 25 aprile, di accoglierli come italiani, come fratelli e come resistenti.

è criticata da molti (anche dall'ONU, per esempio, che non riconosce l'annessione dei territori occupati mentre Israele, ovviamente, la riconosce), allora noi ce la prendiamo con gli ebrei. È una posizione assolutamente inconcepibile: chiunque oggi pensi che si possa organizzare l'odio contro un popolo, contro una razza è fuori dalla grazia di Dio e va fortemente contestato. Anche da questo punto di vista, approvare una

allora è diverso. Anche questa è una garanzia di serietà da parte del Senato della Repubblica. Come il senatore Malan, spero anch'io che finalmente la Camera non debba aggiungere un'altra volta il suo segno e che finalmente questa legge possa venire alla luce. finestra"). Salutiamo studenti e docenti del Liceo linguistico e delle scienze umane «Giovanni Pascoli» di Massa, che stanno assistendo ai nostri lavori. nel libro «Sonderkommando Auschwitz», Shlomo Venezia scrive: «Tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna sempre nello stesso posto... Non si esce mai, per davvero, dal Crematorio». Il Sonderkommando era una squadra speciale, selezionata tra i deportati, con l'incarico di far funzionare la spietata e metodica macchina di sterminio nazista. La moglie di Shlomo mi ha raccontato che suo marito aveva mantenuto anche con lei il riserbo sull'orrore subito, finché il riaffiorare di quei simboli, di quelle parole d'ordine, di quelle idee che avevano generato il mostro dello sterminio nazista fece sì che, nel 1992, decidesse, come altri sopravissuti, che la sua testimonianza poteva e doveva essere un forte antidoto ad ogni follia negazionista. Vorrei dare un piccolo contributo a questo dibattito anche leggendo un breve brano del suo libro: «Dopo che il gas era stato versato, passavano dieci o dodici minuti e non si sentiva più un rumore, più anima viva. (...) Io avevo il compito di tagliare i capelli alle donne. (...) Servivano soprattutto le trecce, facili da tagliare e da trasportare. Dopo il taglio dei capelli e l'estrazione dei denti d'oro, due persone venivano a prendere i corpi per metterli sul montacarichi che li portava al piano terra dell'edificio, verso i forni crematori. I corpi erano tirati fuori e deposti davanti ai forni, due a due. Davanti a ogni muffola tre uomini si occupavano di infornare i cadaveri. I corpi erano deposti su una specie di barella, uno per la testa e uno per i piedi. Due uomini, ai lati della barella, la sollevavano con l'aiuto di un lungo pezzo di legno inserito dal di sotto. Il terzo uomo, di fronte al forno, impugnava i manici e infornava la barella. Doveva fare scivolare i corpi e riprenderla velocemente, prima che il ferro si scaldasse troppo. Gli uomini del Sonderkommando avevano preso l'abitudine di versare dell'acqua sulla barella prima di disporvi i corpi, per evitare che si incollassero al ferro incandescente, altrimenti il lavoro diventava ancora più difficile: bisognava staccare i corpi con una forca e dei pezzi di pelle rimanevano attaccati». Se perdevano tempo sarebbero stati puniti. Certo non possiamo consentire che qualcuno possa negare o banalizzare testimonianze come quella di Shlomo. Sono passati ormai cinque anni da quando ho presentato il primo disegno di legge sul negazionismo, un atto che allora portava - come ha ricordato poc'anzi il collega Malan - come terza firma quella di Rita Levi Montalcini. Ricordo con rammarico che quando, nella difficoltà di far comprendere il valore simbolico di questa norma, facevo notare il peso oggettivo della sua adesione, l'ultimo atto da lei sottoscritto prima della sua morte, purtroppo qualcuno commentava: «Certo, è ebrea». In quel momento, anche qui, c'era chi non riconosceva più la senatrice a vita, il premio Nobel, e vedeva la donna ebrea. Ho deciso oggi di rendere pubblica questa triste circostanza, perché forse in essa si racchiude la verità dei ritardi di questi anni; troppo tempo per portare a compimento un atto semplice, che dà seguito, peraltro, agli impegni presi dal nostro Paese, a partire dalla legge n. 211 del 2000 per l'istituzione del Giorno della memoria, fino all'obbligo al quale ci richiama l'Unione europea dal 2008, con la decisione quadro sul contrasto a talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia attraverso il ricorso agli strumenti del diritto penale. un atto vincolante, in base al quale gli Stati membri hanno l'obbligo di punire l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale,

Paesi come la Francia, la Germania, la Polonia, l'Austria, la Svizzera, il Belgio e i Paesi Bassi già dispongono di norme che identificano il negazionismo come un reato e non possiamo certo dire che questi siano Paesi in cui non esiste libertà d'opinione. Crescono, intanto, preoccupanti organizzazioni neonaziste, come Alba Dorata in Grecia, si rafforza l'estrema destra xenofoba in Ungheria e - come credo sappiamo tutti - in Austria. Proliferano su Internet inaccettabili siti antisemiti e xenofobi, dove si è perfino brindato alla morte di Shlomo Venezia, testimone diretto dello sterminio ad Auschwitz. Ieri era il 25 aprile e nelle nostre piazze, ancora una volta, si sono sentite parole dal cuore e parole di circostanza, ricordando chi, nel sacrificio, ha consentito la nascita della democrazia e della Repubblica. Trovo grave che, ancora oggi, in quei cortei ci sia chi contesta la presenza della brigata ebraica, o che questa venga insultata, come è successo nel corteo di Milano. La storia terribile e gloriosa di chi in quegli anni ha combattuto la dittatura in Italia e il nazismo non si discute. Mi auguro, dunque, che oggi, finalmente, si riesca ad approvare questa norma: un piccolo passo di riparazione del Parlamento italiano che votò nel 1938 le leggi razziste, un atto di contrasto concreto ai fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo e un necessario adeguamento,

che ha coinvolto questa Assemblea in una discussione interessante, svolta su vari fronti, e non solo relativamente al tema in sé a proposito di come inquadrare il tema della punibilità di un atto considerato odioso, distinguendo, allo stesso tempo, l'espressione di una posizione, di un principio, di un convincimento e di un'opinione, per quanto esecrabile e nefanda, da un'azione che possa essere considerata come un reato,

infatti, il tema - sollevato giustamente dentro e fuori dalle Assemblee parlamentari - di una modalità di intervento normativo che

Era un'osservazione legittima, giusta condivisibile perché segnalava il rischio che la nostra azione, volta a punire il negazionismo come un reato configurato a partire a partire dalle sue conseguenze, potesse invece sconfinare nel campo della libertà di opinione. A mio giudizio, abbiamo risolto bene questo problema, evitando di definire il negazionismo come un reato in sé.

della minimizzazione o negazione di crimini feroci contro l'umanità o intere popolazioni,

dall'articolo 3, ossia una posizione negazionista che abbia come conseguenza l'istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza.

agli Stati membri del Consiglio d'Europa di intervenire con l'adozione di misure normative adatte a punire l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale e dei crimini di cui all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale internazionale

ha ritenuto per l'appunto di eliminare questa parola. Io mi auguro - siamo ancora in fase di presentazione degli emendamenti - che il Senato trovi la soluzione adatta per rispettare quel principio. Noi dobbiamo trovare, una volta per tutte, la strada che ci consenta di punire

persino a chi abbia da esprimere delle posizioni assolutamente non condivisibili, che ci appaiono spregevoli ed esecrabili. Dobbiamo accettare

possiamo rischiare che, nel nostro Paese, delle persone vengano punite semplicemente per l'espressione di una loro libera opinione, ma non dobbiamo rischiare neanche l'opposto, e cioè che che discorsi che incitino all'odio, alla violenza o alla discriminazione e siano in grado di produrre fenomeni di questo genere rimangano senza una risposta e vengano intesi nel loro carattere neutro. La decisione quadro del Consiglio d'Europa che citavo prima, che addirittura parla - noi non ci siamo avventurati fino a quel punto - di sanzionare la minimizzazione dei reati di genocidio, dal diritto comunitario e dalla stessa Corte europea dei diritti umani, che ha

di pensiero possono essere considerate libere opinioni e va stabilito il giusto confine fra la libertà di opinione e la produzione di un danno sociale, a partire anche dalla semplice espressione delle proprie opinioni e parole. È un compito molto difficile. Credo che l'equilibrio trovato lo scorso anno in quest'Aula fosse accettabile. Mi auguro che il testo che verrà fuori nei prossimi giorni in quest'Aula

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi per affrontare in seconda lettura il disegno di legge n. 54-C, il quale, per la delicatezza del suo oggetto e delle sensibilità storiche che va a tutelare, è stato caratterizzato da un *iter* ponderato e attento, nonché da una revisione complessiva, nel corso dell'esame, dell'approccio nell'affrontare il fenomeno del negazionismo. Infatti, rispetto al primo testo della Commissione giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del codice penale un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015, aveva inteso ovviare alle criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione e, d'altro canto, alla necessità di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero, di cui si fa garante l'articolo 21 della nostra Costituzione. Tuttavia, come sempre più spesso avviene, anche in questo caso è accaduto che un disegno di legge approvato dalla maggioranza in Senato è stato modificato dalla medesima maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento; e per di più, modificato in maniera incisiva, data l'eliminazione della modifica dell'articolo 414 del codice penale e delle modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Ciò probabilmente è cartina di tornasole su quanto sosteniamo da tempo sulla tenuta complessiva di questa maggioranza e sulla qualità della sua attività legislativa. Eppure, la scelta Eppure, la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. del 1975, rispondeva all'esigenza di circoscrivere la fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare atti di discriminazione ovvero crimini violenti, senza incorrere nel rischio di incidere sulla libera manifestazione del pensiero. A causa delle perplessità suscitate da queste modifiche, emerse nel corso dell'esame, i membri della Commissione giustizia del Senato e, *in primis*, la relatrice hanno convenuto che il testo licenziato in prima lettura fosse più corretto, cosa che ha portato al recepimento delle proposte emendative, comprese quelle del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, che ripristinano quasi *in toto* i contenuti del testo trattato al Senato. È evidente, quindi, che non perverremo oggi all'approvazione definitiva di questo disegno di legge. Sul negazionismo anche il nostro Paese dovrebbe assumere una posizione netta, così come hanno fatto gli altri Stati europei. Il fenomeno del negazionismo si è manifestato con portata e in misura diversa a seconda dei Paesi europei e, attualmente, è punito espressamente in Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna, Portogallo e Svizzera. Pertanto, così come in molte altre situazioni che si sono verificate nel corso di questo Governo, sarebbe opportuno decidere definitivamente se si vuole agire affidando a una norma la disciplina della questione, in tal caso farlo al più presto, in maniera compatta e decisa; oppure se non si voglia affrontare il problema da un'altra prospettiva, eminentemente culturale. Come scrisse Timothy Garton Ash, saggista e docente dell'università di Oxford: «La negazione dell'Olocausto va combattuta nelle scuole, nelle università, sui nostri *media*, non nelle stazioni di polizia e in tribunale». Il negazionismo è una vergogna ed è un orrore da contrastare sempre, compiendo tutti gli sforzi possibili per far vivere e per trasmettere la memoria della Shoah; lo è tanto di più oggi, di fronte all'intreccio sempre più temibile e talvolta sanguinoso tra i vecchi e mai sopiti germi di antisemitismo e inediti fenomeni di odio globale, a cominciare dall'islamismo È emblematica la sciocca reazione di una frangia dell'antagonismo ieri, 25 aprile, a Milano, durante il passaggio della brigata ebraica. Da questo punto di vista, sembra mortificante per le coscienze libere e democratiche che, per affermare una verità di assoluta evidenza, cioè il carattere raccapricciante, odioso e unico della Shoah, sia necessario ricorrere a una norma di legge. Inoltre, stabilire legislativamente una verità storica di Stato rischia di offrire un alibi all'incapacità che abbiamo tutti come corpo sociale, costituito dalla scuola, dal sistema educativo, dalla famiglia e dalla società civile, di contrastare il negazionismo sull'unico terreno appropriato: il terreno dell'educazione, dell'informazione, della divulgazione culturale. Educazione, corretta informazione e studio della storia dovrebbero, pertanto, costituire gli anticorpi per contrastare quella scellerata scelta di una parte dell'umanità di negare il crimine più efferato che mente umana abbia concepito: la distruzione di massa di sei milioni di ebrei. Pertanto, avendo preso coscienza di questi due diversi e possibili approcci (quello legale e quello educativo) in una difficile mediazione individuale e collettiva delle esperienze e delle sensibilità culturali e politiche, se il più efficace per il nostro Paese appare essere quello in cui prevale l'aspetto punitivo e sanzionatorio più che educativo, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà in favore di uno strumento che è comunque portatore di una memoria storica che deve essere sempre tutelata, in quanto espressione di una irrinunciabile religione civile che tanto ci insegna, tanto ci esorta, tanto ci impone responsabilmente di ricordare.

dichiara la difficoltà di prevedere una norma comunque difficile, ma di sicuro evidenzia un grosso problema di natura politica. A questo punto il prevedere o meno questa

posso ricordare uno dei grandi fenomeni di strabismo storico. Nel testo si parla della Shoah, dell'Olocausto,

stessi: noi siamo fatti di storia e il nostro futuro dipende dalla nostra storia. È quindi vero che, per certi versi, negare è una menzogna, ma chi dice che la menzogna debba necessariamente diventare reato?

questo era il tema delle foibe, negato per una questione politica. Ora ci troviamo a parlare di un'ipotesi che, tra l'altro, va a inserirsi in una legge già di per sé

commette il reato: che cosa significa propagandare idee fondate sulla discriminazione? Già l'incitamento

di propaganda o dell'incitamento all'odio razziale, esso deve avere una portata nociva per diventare reato, deve essere una condotta di per sé pericolosa. Pertanto

per ragionare se sia veramente necessario far passare attraverso una previsione normativa quello che dovrebbe essere nient'altro che un intervento di natura culturale.

ho una qualche difficoltà a intervenire su un provvedimento di cui non conosco gli emendamenti che saranno presentati domani entro le ore 13. Con un'approssimazione dovuta a queste ragioni e anche a un mio impedimento personale,

Naturalmente questo provvedimento non ha nulla a che fare con il negazionismo, neanche lontanamente. Abbiamo sentito storici in Commissione dividersi: sostanzialmente l'80 ha negato la necessità di una legge che trattasse il problema del negazionismo in generale; una minoranza invece ha detto ‑ ed ero d'accordo anch'io ‑ che, davanti a tragedie della storia come l'Olocausto a genocidi programmati come quelli del secolo scorso, una legge che colpisca specificatamente quella - spero irripetibile - pagina nera della storia dell'umanità poteva essere anche fatta.

Poi, viceversa si è detto di limitarlo soltanto alle sentenze delle corti internazionali e, se non erro, nel testo pervenuto in Aula sono sparite anche le corti internazionali. Adesso vi leggo alcune delle fattispecie per cui uno potrebbe essere denunciato e avere anche l'aggravante prevista dalla legge. Per esempio, crimine di guerra violare la dignità personale, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti, e distruggere o confiscare i beni dell'avversario. Il crimine di guerra è la Il crimine di guerra è la distruzione o l'appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta su larga scala illegalmente o arbitrariamente; è costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle Forze armate di una potenza nemica; è la deportazione, un trasferimento o detenzione illegale; è una cattura di ostaggi. E si continua così per quattro pagine.

modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre

dice: «in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale». Scusate, cosa c'entra il negazionismo?

che è stata costruita, purtroppo, su dati religiosi, etnici, razziali: è così, perché l'etnia nelle guerre balcaniche ha avuto

un qualcosa che limiti la responsabilità di una delle parti in lotta rispetto alle altre, rispetto a migliaia di casi, perché qualcuno a cui non piace ciò che stai dicendo pubblicamente ti denuncia? Si dice di stare

almeno per correggere alcune delle forzature più evidenti di questo disegno di legge, magari limitandolo soltanto al genocidio, che è già qualcosa, ma sicuramente non alle decina di migliaia di casi di cui si interessa e attraverso cui si va a colpire un principio fondamentale come quello di ricerca, di studio e anche il sostegno di tesi che possono essere in contrasto con quelle di qualche organismo internazionale.

a esprimere argomenti sensati e forti in merito al provvedimento in esame, perché a me sembra di assistere a un gioco delle parti a un gioco delle parti promosso dalla stessa maggioranza, che ci costringe ad esaminare in seconda lettura - quindi questa è la terza volta che le Camere affrontano lo stesso provvedimento - un testo che per volontà stessa della maggioranza, come se fosse bicefala o schizofrenica, è stato sottoposto a revisione tra Camera e Senato. Questo accade perché che interviene su un problema i cui contorni non sono particolarmente perimetrati. Infatti, come è stato e diversi colleghi che mi hanno preceduto l'hanno rimarcato, se da un lato c'è una sorta di imperativo morale ad evitare di dire falsità, è altrettanto vero che trasferire tale imperativo morale nel codice penale, facendone un reato, comporterebbe, per esempio per chi è qui dentro

perché se un provvedimento fa la navetta così frequentemente, evidentemente è il metodo è il metodo che è sbagliato. Io mi domando se piuttosto che il metodo non sia sbagliato il manovratore,

con i loro omologhi della Camera per capire quale sia il testo su cui si deve lavorare. Detto questo, intervengo un po' più nello specifico. Come diceva giustamente il senatore Giovanardi, di fatto alla fine la montagna ha partorito un topolino perché si interviene producendo semplicemente un'aggravante un'aggravante per un'ipotesi di reato già prevista da un'altra legge. Ora, si deve entrare nel merito dei reati d'opinione e, in particolar modo, bisognerebbe domandarsi cosa sia l'istigazione a delinquere perché questo è il vero problema. Quand'è che io istigo ma soprattutto, domandiamoci, chi è che può essere istigato da qualcuno che sta dicendo scemenze, scemenze, ovvie falsità? Probabilmente chi può essere oggetto di istigazione è un soggetto facilmente manipolabile, facilmente condizionabile e nell'epoca in cui domina la scena lo *storytelling* renziano forse vi è necessità di intervenire perché ormai la storia è distinta dalla storiografia da chi lo sa; ma in un momento in cui tutto è miscelato, tutto è mischiato, bisogna fare attenzione, appunto, alla narrazione, allo *storytelling*, quasi dovendo imparare a distinguere una serie televisiva dalla realtà. Questo, forse, è lo

a tramutare in legge altre parole che tutti hanno concesso essere sensate. Mi riferisco alle dichiarazioni del procuratore antimafia Roberti, secondo il quale tutti quanti, a parole, in ambito politico, riconoscono cosa si debba fare, salvo poi essere pochissimi quelli che davvero si battono in queste Aule per introdurre norme che penalizzino effettivamente l'associazione a delinquere, la corruzione, l'evasione fiscale. Queste sono, ad esempio, tre brutte bestie da combattere e su cui questo Parlamento sta facendo ben poco. Se spendessimo la metà del tempo che abbiamo speso per esaminare questo per produrre atti normativi che gli stessi magistrati attendono da tempo immemorabile, noi avremmo fatto un favore all'Italia e un favore alla alla cultura e all'intelligenza critica. Recuperando risorse, avremmo impedito alle persone di essere gettate nel cono d'ombra dell'ignoranza; perché è soltanto la dimensione dell'ignoranza quella in cui può sapientemente pescare chi vuole predicare Mi scusi, ma era era la passione. Si tratta di scemenze, di assurdità, quelle per cui si può spendere un argomento assolutamente destituito di fondatezza storica e scientifica per istigare qualcuno a compiere ciò che mai e poi mai deve essere commesso. E uno Stato che sia veramente civile e democratico investe in cultura, perché attraverso la cultura si previene il reato, e non tanto in repressione perché è soltanto l'ignoranza ciò che lo concede.

intervengo per segnalare una cosa che a me pare degna di nota e che riguarda la vicenda della

Il presidente di quella associazione, Giorgina Secci, ha fatto per sedici giorni consecutivi uno sciopero della fame prima che qualcuno si interessasse alla sua questione. Giorgina Secci richiede che venga istituito un punto di guardia medica per il proprio Comune, perché Urzulei, un paese di 1.300 anime, sta sopra le montagne della Sardegna, al centro della Sardegna, in una condizione di isolamento aggiuntiva a quella che tutti quanti i Comuni della Sardegna subiscono per essere Comuni di un'isola. Un paese nel quale le 1.300 anime non hanno un medico, non hanno un punto di guardia medica, dove mancano tanti altri servizi che pure sono pure sono erogati in tante altre realtà. Giorgina Secci fa lo sciopero della fame per richiedere attenzione e mi pareva giusto segnalare questa vicenda come emblematica della condizione di isolamento nella quale si sentono le nostre zone interne, vittime spesso anche di difficoltà e crisi sociali ed economiche acute. Urzulei è un paese di antica storia, abitato già in epoca nuragica, inserito in uno splendido paesaggio montano, ma lontano. Noi abbiamo un dovere verso ogni uomo e ogni donna che sceglie di vivere nei nostri piccoli paesi dell'interno: quello di ringraziarli per la loro lotta concreta e quotidiana contro lo spopolamento della terra di Sardegna. E penso anche ad altre terre, signor Presidente, come quelle delle sue Regioni, quelle montane, montane, che subiscono e sono vittime dell'isolamento e spesso della trascuratezza delle istituzioni pubbliche; quelle che non stanno dentro i criteri dei costi *standard*. Quelle che meritano - per il fatto stesso che vengono fatte salve una cultura, una

ho potuto direttamente prendere atto di una situazione paradossale: c'è una struttura privata, messa a disposizione della Croce Rossa, che ospita, ormai da più di nove mesi,

fino ad arrivare a pretendere di essere condotti dal prefetto, il quale ha accolto la loro richiesta di audizione. Premesso che, se ci troviamo in un Paese in cui chiunque inscena una manifestazione

per cento non sarà riconosciuto come tale, è ormai ospite da parecchi mesi, a spese della collettività tradatese, che paga le tasse. In un anno, questi cittadini stranieri costeranno più di un milione di euro: il costo si stima infatti intorno al milione o al milione e mezzo

La situazione non può essere gestita così. Continuiamo a chiedere al Governo di costruire strutture veloci per definire lo *status* giuridico: chi ha diritto a restare, perché rifugiato, deve veder riconosciuto il proprio diritto entro pochi giorni. Chi non ne ha diritto, deve essere rispedito al Paese di provenienza, perché non possono crearsi situazioni di tensione nelle nostre comunità, per di più con aspetti diseducativi, visto che queste persone sono in giro tutto il giorno a bighellonare, forniti dei migliori telefonini,

a sostenere questo sistema di accoglienza insensato e, aggiungo anche, signor Presidente, in maniera addirittura paradossale, portando questi stranieri clandestini richiedenti asilo in giro per le manifestazioni pubbliche, utilizzandoli come per dare sostegno e clamore alle iniziative dell'amministrazione. Non ci siamo: siamo il Paese che sta invertendo il rapporto tra i cittadini e gli ospiti. Gli ospiti, se hanno diritto, siano ospitati, altrimenti siano rinviati a casa e i cittadini siano rispettati per le tasse e la fatica che fanno ad essere cittadini fino in fondo.